di voci false. Chi ha partecipato con me all'assemblea del Gruppo e ha ascoltato l'intervento del Capogruppo ha preso atto che è stata svolta una analisi molto lucida su quanto sta avvenendo in Parlamento e anche alla Presidenza del Consiglio. Stiamo assistendo ad un'autentica compravendita del consenso parlamentare: ne abbiamo preso atto. Abbiamo anche preso atto che questo Governo non governa: quindi, in realtà questo

la Commissione bilancio si è riunita ieri su suo mandato, ed è tornata ad esaminare il problema degli effetti rispettivamente sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento dell'approvazione in Commissione dell'emendamento 3.2000. Ferme restando le posizioni della maggioranza e dell'opposizione sia sulla ricevibilità, come nota tecnica prevista dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, della nota consegnata in Commissione dal sottosegretario Sartor in risposta alla richiesta di nota tecnica sull'emendamento 3.2000 avanzata al Ministero dell'economia dalla Commissione stessa,

per la competenza, cioè ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ciò che è ovvio per tutti, maggioranza e opposizione, ma anche per la cassa gli effetti negativi sull'indebitamento, indotti dalla particolare forma di copertura adottata per l'emendamento in questione, l'intera Commissione ha potuto con soddisfazione prendere atto dell'avvenuta presentazione, da parte del Governo, di un emendamento che figura al nostro esame come emendamento 14.800, che compensa perfettamente, per gli anni di riferimento, gli effetti negativi sull'indebitamento quantificati dall'aggiornamento, dopo l'esame in Commissione, dell'allegato 7, debitamente vistato dal Ministro dell'economia, secondo le procedure tradizionali. Naturalmente la Commissione la Commissione non si è soffermata, anzi non ha affatto discusso sul giudizio di merito, cioè sul giudizio politico delle scelte operate dal Governo nell'emendamento in questione. Questo giudizio è infatti affidato perfettamente all'Aula come su tutti gli altri emendamenti.

a valutare - e lo ha fatto positivamente - la capacità dell'emendamento sul piano strettamente tecnico‑formale di superare le obiezioni mosse in merito ai caratteri e agli effetti della copertura dell'emendamento 3.2000. Preso atto che l'emendamento compensa gli effetti negativi sull'indebitamento fatti emergere, anche sotto il profilo cognitivo, dall'allegato 7, come attestato dal Ministero dell'economia, e lo fa secondo la prassi di certificazione della regolarità delle coperture adottata nella procedura interna alle decisioni del Ministero dell'economia, la Commissione mi ha incaricato di riferire in questo senso in Aula. Colgo l'occasione, signor Presidente, per tornare a sollecitare l'esame da parte della Giunta per il Regolamento delle proposte, avanzate ormai da mesi, al termine della discussione in Commissione bilancio sulle procedure della sessione di bilancio.

ma è indispensabile non disperdere questo capitale di consenso e metterlo immediatamente a frutto attraverso le conseguenti e coerenti modifiche del Regolamento. Signor Presidente, termino facendole notare che anche la discussione, a mio avviso trasparente e qualitativamente importante, che abbiamo fatto a proposito della questione che - credo - con questa mattina si chiude, si chiude, deriva da alcune modificazioni di prassi adottate consensualmente (centro-sinistra e centro-destra) in Commissione bilancio, e fatte proprie dal Presidente al fine di interpretarle sotto il profilo della conduzione dei lavori, che hanno bisogno di essere sancite. In particolare: la regola che vuole che il Governo e il relatore di maggioranza presentino i loro emendamenti contemporaneamente ai parlamentari e non possano presentarne successivamente su nuovi argomenti; la regola che vuole che gli emendamenti del relatore siano corredati da relazione tecnica esattamente come gli emendamenti del Governo (abbiamo adottato questa prassi ma non è scritto nel Regolamento); aggiungo persino la regola che vuole che sugli emendamenti parlamentari di maggiore rilievo, su cui relatore e Governo esprimono un consenso ed una approvazione, vengano sottoposti immediatamente all'obbligo di presentazione della relazione tecnica; la regola che vuole che i lavori della Commissione bilancio si concludano in modo tale che sia possibile aggiornare l'allegato 7 e informare l'Aula degli effetti complessivi, certificati dal Ministero dell'economia, degli emendamenti che sono stati approvati in Commissione in maniera tale che le decisioni siano prese sempre con perfetta cognizione di causa. Ecco, queste regole fondamentali, che abbiamo adottato in via di fatto,

ad alcune fanfaluche affermate in quest'Aula oltre che ad arrampicate sui vetri per dimostrare l'indimostrabile e poi la realtà è stata che il Governo ha dovuto presentare un emendamento per correggere la norma scoperta con la quale in Commissione si era affrontata la questione dei *ticket*. Ovviamente la maggioranza ha dovuto difendere il fatto che l'emendamento fosse ammissibile. A nostro avviso non lo era, tanto è vero che non lo era, tanto è vero che il principio di non contraddizione è stato contraddetto, perché affermandosi che non era ammissibile l'emendamento e che non necessitava di copertura, alla fine il Governo ha dovuto porvi rimedio presentando un emendamento di copertura. Concludo ringraziandola, signor Presidente, per aver avuto ieri la sensibilità di sospendere la seduta prima dell'esame dell'articolo 3 in modo da consentire la predisposizione di un emendamento che modificasse anche l'articolo 3, senza il quale tutto il procedimento sarebbe rimasto viziato. Resta - e con questo concordo con il presidente della 5a Commissione Morando - il fatto che gli emendamenti vanno coperti anche con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento che

d'ora in poi, tutti gli emendamenti governativi e del relatore dovranno essere dotati di adeguata relazione tecnica, il che mi sembra, alla fine della vicenda e malgrado lo scivolone del Governo e della maggioranza,

La relazione tecnica, come sappiamo, è competenza del Ministero dell'economia. Ci sono state, soprattutto nella discussione in Commissione, delle divergenze con la Ragioneria generale dello Stato, tuttavia tali divergenze - è inutile negarlo - sono state evidenziate dallo stesso Governo tramite l'intervento del sottosegretario Sartor. Questa è la pura verità: non c'è stato uno scontro all'interno del Ministero dell'economia; ci sono state delle valutazioni diverse evidenziate in modo preciso e trasparente da parte del sottosegretario Sartor. Chi è il responsabile della relazione tecnica? È il Governo, in questo caso il Ministero dell'economia. Io ritengo che il Governo abbia garantito correttezza e trasparenza; anzi, penso che se non avessimo adottato quella procedura, cioè quella di prevedere che anche il Governo e il relatore presentassero i loro emendamenti nei tempi previsti per i Gruppi parlamentari e per i singoli senatori, e che questi emendamenti fossero accompagnati da relazione tecnica, questa discussione - che, ripeto, garantisce correttezza e trasparenza - non ci sarebbe stata; non ci sarebbe stato questo confronto tra la maggioranza e l'opposizione. Quindi ringrazio

credo che sia un qualcosa in più che viene offerto alla nostra discussione, che ci garantisce di più rispetto ai problemi che stiamo affrontando. È una posizione ineccepibile dal punto di vista tecnico; formalmente - ripeto - un qualcosa in più rispetto a quanto era dovuto. Per quale Perché sul fabbisogno non c'era necessità di alcuna correzione; siamo comunque sotto il 3 per cento, siamo in linea con le previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria. Infine, la questione della trasparenza e del controllo.

bilancio la decisione unanime - questo va ricordato - di stabilire regole nuove nell'esame dei documenti di bilancio. Abbiamo fatto un buon servizio al Parlamento; non lo abbiamo fatto su proposta dell'opposizione. Personalmente ritengo che il servizio sia stato soprattutto a favore della maggioranza, perché non si è più verificato in questa sessione di bilancio quello che accadeva negli anni passati, sia nella scorsa legislatura che in quella precedente, quando il Governo poteva fare quello che voleva, presentava i maxiemendamenti senza alcun controllo e poi il Parlamento veniva chiamato *ex post* a garantire una copertura formale. Questo non è più avvenuto. Credo che tutto ciò sia una garanzia per tutti, per l'opposizione ma anche per la maggioranza, perché in questo modo può esercitare meglio il proprio controllo sugli atti del Governo. *(Applausi

perfezionamento della norma di copertura a valere sull'indebitamento. Ma non c'è dubbio che la copertura, con riferimento al saldo netto da finanziare, era corretta, da finanziare, era corretta, che l'emendamento era perfettamente ammissibile e che i comportamenti del Presidente della Commissione e del relatore, nella gestione dello stesso, sono stati assolutamente ineccepibili. questo rimanga agli atti del Senato perché è l'elemento fondamentale, centrale della nostra discussione. Chi sostiene l'inammissibilità dell'emendamento dice una cosa non vera. La seconda osservazione è altrettanto breve ed è la seguente. L'episodio ha per certi versi un aspetto virtuoso, nel senso che evidenzia come il comportamento

Il presidente Morando ha ricordato la necessità di sancire, anche dal punto di vista regolamentare, alcune norme che abbiamo già applicato nel corso del dibattito su questa l'obbligo per il relatore e per il Governo di presentare gli emendamenti nello stesso tempo prescritto per i parlamentari, l'obbligo della relazione tecnica per gli emendamenti del relatore e per quelli importanti che il Governo intende accettare. accettare. Abbiamo già concretamente dimostrato come si possa lavorare sulla finanziaria in modo trasparente, avendo la certezza dei numeri e dei risultati. Non possiamo accettare che passi l'idea di una finanziaria poco chiara,

cui abbiamo lavorato anche in Commissione bilancio su questo tema. Signor Presidente, condivido quanto ha affermato il collega Morando. È importante che le regole che ci siamo dati autonomamente

Ora i colleghi hanno cercato di indorare la pillola - per carità - ma il dato di fatto è che, grazie anche alla sua esposizione e a un suo senso della misura,

perché hanno evitato che si creasse in qualche modo un precedente che poteva poi valere anche nella prossima legislatura, nella quale ovviamente speriamo che la compagine governativa sia differente. fatto, una volta che si mette una regola e che il Governo, in quanto autorità amministrativa, è "obbligato" dalla sovranità popolare del Parlamento a comportarsi in un determinato modo, ossia

La sostanza è che si è dovuto ricorrere ad una nuova copertura. Ora la copertura è stata pubblicata, la vedremo, Presidente, e ne discuteremo nel momento opportuno.

è un aggregato statistico, convenzionabile dall'EUROSTAT, come se negli ultimi 15 anni tutti i Paesi europei, Italia in testa, non abbiano dovuto seguire purtroppo, quasi mese per mese, l'andamento di questo importante aggregato di finanza pubblica. È chiaro che i colleghi della maggioranza hanno difficoltà, perché si trovano di fronte ad un Governo spesso pasticcione, qualche volta imbroglione nei conti. La dimostrazione di ciò è appunto l'emendamento di cui

Probabilmente, dovremo prepararci tutti, per il prossimo anno, a vedere spuntare altri 13-14 miliardi di euro. È questo il punto, signor Presidente, non tanto l'aggiustamento dovuto, da parte del Governo, per 350 milioni di euro, che vengono sistemati stamattina con l'emendamento 14.800. Il punto è l'incertezza, la fragilità, la manipolazione manipolazione dei conti pubblici che il Governo ha esercitato fin dal suo primo giorno, quando annunciò al Paese che il *deficit* pubblico l'anno scorso sarebbe salito oltre il 5 per cento del PIL, fuori da ogni grazia di Dio, in realtà - come sappiamo - è stato ed era abbondantemente sotto il 3 per cento, al 2,3 per cento. La verità è che l'azione di questo Governo ha raddoppiato il *deficit*

una copertura credibile, anche perché la stessa Ragioneria dello Stato ci confortava con il suo diniego, rifiutandosi di riconoscerla e di apporre la firma. avete ostinatamente sostenuto una tesi opposta, accettando un emendamento che doveva ritenersi inammissibile.

Collega Ripamonti, un mio amico che cadde dalla bicicletta disse: qui dovevo scendere! Questa mattina lei ha fatto lo stesso lo stesso dicendo che siete stati bravi e trasparenti perché avete messo i conti a posto. No! Siete stati obbligatoriamente trasparenti perché, grazie alla ferma opposizione del centro-destra, siete stati costretti

dobbiamo, però, positivamente dire che il presidente Morando e la maggioranza della Commissione bilancio hanno preso coscienza di questo errore ed hanno promesso che nel futuro non si ripeteranno situazioni di questo tipo. Ne prendiamo atto e saremo rigidi ed attenti perché non si ripetano.

Presidente, colleghi senatori, partiamo da un fatto: eravamo di fronte,

e ci fu illustrata dal sottosegretario delegato alla finanziaria, professor Sartor. Si è trattato quindi di una tempesta in un bicchiere d'acqua. La copertura c'era ed è indirettamente confermata dall'emendamento tecnico, senatore Baldassarri, che lei ha citato, di

sulla Tabella A siamo di fronte ad una compensazione di basso valore economico. Lo si poteva fare anche alla fine quando, come in ogni finanziaria (lo sanno meglio di me i senatori che ne hanno fatte di più), si prende atto degli eventuali scostamenti, frutto degli impegni aumentati a causa di emendamenti approvati. Abbiamo qui, con la relazione citata ieri, il dato dei saldi aggiornati rispetto agli emendamenti votati in Commissione ma, come è noto, il bilancio prende atto, alla fine della discussione parlamentare, dei saldi.

e sale solo nel 2009 e nel 2010. Presidente Marini, colleghi senatori, il lavoro del Parlamento nella sua Commissione bilancio ha ridotto in maniera positiva il saldo per il 2008. Altro che aumento delle spese e dell'indebitamento! È per questo che vorrei concludere le mie brevi note esprimendo piena solidarietà e consenso al presidente della Commissione,

nella sua prima stesura. E lo si è risolto, dimostrando che è bene che Parlamento e Governo interloquiscano nell'interesse del Paese. Presidente, non intervengo nel merito perché l'ha già fatto il collega Baldassarri, però, dopo quanto è accaduto ieri e anche dopo le mie insistenze, rivolte proprio a lei perché prendesse una decisione, come le competeva, desidero ringraziarla. Infatti ieri, nella Conferenza dei Capigruppo, lei ha fatto una scelta di buonsenso, che questa mattina questa mattina ha dato i suoi frutti. Si evince in modo chiaro che avevamo ragione a sostenere che non c'era copertura la maggioranza ha fatto ammenda di ciò, anche con un comportamento un po' strano, perché questa notte in Commissione è arrivato il Ragioniere generale dello Stato per trovare una soluzione. Desidero però darle atto che il suo buonsenso ha riportato a verità

Presidente, poiché il collega Ciccanti ha molto opportunamente precisato in che settore sono intervenute le modifiche, desidero che i colleghi sappiano, perché questo è oggetto di polemica molto seria,

La copertura comprende ora anche i fondi comunitari, che, come tutti sappiamo, sono prevalentemente quelli degli enti locali dell'Obiettivo 1, quindi riguardano soprattutto il Mezzogiorno. La politica antimeridionalistica del Governo risulta rafforzata in modo clamoroso.

È bene che si sappia che questa finanziaria contiene un nuovo attacco al Mezzogiorno ed una smentita ufficiale del ministro Padoa-Schioppa. Da questo punto di vista la si può anche approvare, ma occorre capire che su queste due questioni noi non riteniamo conclusa la vicenda.

molto più importante e molto più grande, quella dei distretti industriali, che esprimono le quattro eccellenze manifatturiere: l'agroalimentare, l'abbigliamento-moda, l'arredo casa, l'automazione meccanica.

L'abbigliamento-moda e l'arredo casa hanno generato un valore aggiunto pari a 42 miliardi di euro, superiore a quello dell'industria tedesca.

a favorire la piccola industria e l'artigianato. In particolare, l'emendamento 3.1 tende a sopprimere la detrazione di imposta

o noi riconosciamo le detrazioni IRAP per lavoratore, e questa è la linea che ha scelto il Governo ed è la linea dei grandi gruppi imprenditoriali di Confindustria (che non criminalizziamo, per carità, per cento dei soldi ai grandi gruppi industriali), oppure stabiliamo una base, cioè una deduzione fissa dell'IRAP non per singolo lavoratore,

per ricordare che l'articolo 3 è uno degli articoli fondamentali di questa legge finanziaria ed uno di quelli che i cittadini cominceranno ad assaporare - lo dico in maniera ironica, ovviamente - a partire dal 1° gennaio. Sotto il profilo politico, questo è l'articolo più straordinariamente ipocrita della legge finanziaria. Perché? Si presenta bene, con una riduzione delle aliquote, con l'idea di una riduzione del carico fiscale in genere, però, incredibilmente, non comporta diminuzione delle entrate dello Stato.

e avviene in modo da penalizzare due tipologie di imprese in particolare: la grande platea delle piccole e medie imprese, naturalmente, e quelle che hanno un tasso di

inferiore a quello delle imprese più grandi. Ed allora, che cosa fa questo straordinario articolo? Tassa una quota degli interessi deducibili, con la straordinaria

Come potete capire, diventerà difficile per un'impresa sostenere un carico di questo tipo. È vero che, come spesso usano fare Governo e maggioranza, questa normativa è condita di parole inglesi straordinarie, come *thin capitalization* o altre, ma io preferisco sempre tradurre in italiano le parole inglesi così sono, almeno per me, più facilmente comprensibili. Questo significa che si cerca forzosamente di capitalizzare le imprese, come se queste non volessero farlo, e quindi si annida, in queste norme, oltre al danno di cui ho parlato prima, l'intento dirigista a cui questo Governo non sa rinunciare in nessun modo. In sostanza il Governo disegna un tipo d'impresa per lui perfetta e chiede che tutti gli altri vi si adeguino. Questo schema di ragionamento era proprio delle pianificazioni centralizzate ed è stato drammaticamente battuto dalla storia ormai in tutto il mondo, mentre qui lo stiamo riproponendo.

l'innovazione tecnologica ma si disincentiva la possibilità per l'impresa di recuperare produttività attraverso l'acquisto di macchinari.

Siccome, signor Presidente, un indizio non fa mai prova, per essere certi che sia questo l'indirizzo del Governo, vi è un'ulteriore norma nell'articolo 3 che conferma quanto ho detto: il *leasing*, che è un altro degli strumenti che le imprese utilizzano proprio per i macchinari ad alta obsolescenza, perché consente loro la restituzione anticipata del bene e l'acquisto di un altro pagando sempre un certo canone, viene penalizzato,

per le imprese e invece qui lo si irrigidisce appositamente, sempre con le stesse conseguenze. Infatti un *leasing* più lungo non può che significare l'emersione di nuova base di reddito.

artificiosamente si allarga la base imponibile, immettendo, nella base imponibile tassabile, una quantità di reddito non effettivo, così contravvenendo al principio generale della effettività del reddito su cui l'imprenditore

elevato a reddito solo per delle imposizioni della legge. Signor Presidente, non ci siamo: questo è uno degli articoli che gli italiani subiranno in maniera drammatica a partire da gennaio e che, insieme a quelli dell'anno scorso scorso per l'economia italiana, in questo clima che si preannuncia leggermente tempestoso (dico leggermente sempre in chiave ironica), produrranno in futuro norme i cui effetti si faranno sentire in maniera pesante sull'aumento della produttività in particolare e del prodotto interno lordo in generale. Faccio solo un altro esempio, signor Presidente. Ho chiesto informazioni alla maggioranza, ed ho trovato consenso sia dal Governo che dalla maggioranza, su un particolare comma che è veramente offensivo. verità, questa finanziaria, mi consenta solo una battuta, fa un esercizio simpatico: sopprime, modifica o integra i commi della finanziaria scorsa, diverse decine se non qualche centinaio di commi sono modificati, ma qualcuno lo fa in maniera negativa. Si pensi al comma 18 dell'articolo 3. Signor Presidente,

Il che significa che le imprese avevano fatto degli investimenti - siamo alla fine del 2007 - già dal 2006 o dall'inizio del 2007, per i quali avevano utilizzato, si accingevano ad utilizzare o avrebbero utilizzato nel 2008 tale credito, grazie ad una legge in vigore. Con il comma 18 si dice: «Beh, signori, abbiamo scherzato, non c'è più il credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno», che già lo hanno

siamo ad una legge che è un *vulnus* allo statuto dei diritti del contribuente; è retroattiva e le norme fiscali non devono esserlo, se non in casi eccezionali e questo non si configura come uno di essi; si abbatte su imprese che hanno realizzato investimenti sapendo di aver diritto ad un credito d'imposta, e poi non lo si fa più; infine si mortificano, ancora una volta, le energie migliori del Mezzogiorno d'Italia, di coloro cioè che intraprendono, che si muovono per dare benessere a quella zona d'Italia, che cercano in tutti i modi di entrare nel mercato competitivo che attualmente si trovano a dover affrontare. Con queste ragioni, signor Presidente, ritengo illustrati tutti i nostri emendamenti all'articolo 3.

clamorosi che penalizzano la struttura portante della nostra economia fondata sulle piccole imprese. Con questa operazione di finanza pubblica voi date un colpo mortale al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. La nostra azione è, allora, andata in questo senso. Il senatore Azzollini ha poco fa richiamato l'attenzione sull'azione che operate attraverso il calcolo degli interessi. Con tale operazione colpite in modo decisivo tutte le piccole e medie imprese, quelle che sono più indebitate, che sono nella fase dello *startup*, che hanno fatto investimenti, che operano con la pubblica amministrazione e con le commesse pubbliche, tutte quelle che soffrono per un sistema che naturalmente ha bisogno di correzioni e non di queste scelte che voi fate. Voi colpite le aziende nel momento in cui operano scelte d'investimento e, quindi, attraverso una violazione clamorosa ancora dello statuto del contribuente. È chiaro che poi

si va a colpire un settore che muove l'economia. Come potete poi lamentarvi che i fondi vadano in Lussemburgo ed in Irlanda, dove c'è un ambiente giuridico più favorevole? Lo stesso accadrà anche per i fondi di

il ministro Bersani si è dimostrato favorevole a rilanciare la rottamazione. Io mi stupisco che il Gruppo dei Verdi non abbia colto questa opportunità. Si fanno paladini della lotta all'inquinamento, ma poi non conducono battaglie coerenti per portare l'inquinamento ad

Oltremodo, la rottamazione ha determinato un saldo positivo ai fini fiscali, perché ha provocato un maggiore gettito anche rispetto al presunto costo ipotizzato nella precedente finanziaria. Io mi auguro che su questo aspetto attenzione da parte di questa'Aula. La questione più rilevante, però, è quella da noi posta rispetto alla necessità di ridurre la pressione fiscale nei confronti delle micro e piccole imprese più strutturate, che sono escluse sia dai benefici dai benefici connessi con il nuovo regime dei minimi che dalle riduzioni di imposta dovute alla riduzione dell'aliquota IRES. Noi proponiamo un innalzamento della deduzione forfetaria IRAP, dagli attuali 8.000 sino a 10.000 euro. Anche il senatore Angius si è fatto carico di tale problema e io mi auguro che su questo punto, così importante e rilevante per le micro e piccole imprese, vi sia uno scatto di orgoglio, che superi i vincoli di maggioranza e possa determinare un voto d'Aula che non vada incontro agli interessi delle forze politiche ma della struttura portante della nostra economia. *(Applausi

Per sostenere lo sviluppo economico, il fisco può costruire un ambiente di vantaggio intorno alle imprese impegnate a compiere un salto di crescita per investimento, per ricerca in nuovi prodotti, per fusione, per il rafforzamento patrimoniale e per forma giuridica; "salti di crescita" sono portatrici di esternalità positive. Queste ultime devono trovare riconoscimento in un sistema fiscale che affianchi al prelievo ordinario un prelievo agevolato atto a premiare percorsi aziendali meritori. Siffatto sistema di premialità deve essere impostato in chiave dinamica, agevolando le imprese che compiono scelte non inerziali e con l'esplicito intento di modificare, anche radicalmente, la propria configurazione di mercato. Il disposto dell'articolo 3 della legge finanziaria, che stiamo oggi discutendo, non va interamente in questa direzione. Ciò che si propone è un abbassamento generalizzato delle aliquote IRES, a fronte di un allargamento della base imponibile. Dunque, sebbene le proposte contenute nella legge finanziaria beneficino le imprese aventi una struttura di bilancio robusta, tali proposte non aiutano a costruire un vero e proprio sistema premiale per almeno due ragioni. In primo luogo, i benefici vengono distribuiti in base alla composizione attuale del sistema produttivo, senza prevedere premi per quanti si impegnano in salti di crescita. Ossia, il provvedimento all'articolo 3 manca di una visione dinamica. In secondo luogo, un sistema premiale non si costruisce penalizzando monetariamente le imprese più deboli. Queste devono essere aiutate a crescere, non richieste di finanziare surrettiziamente, attraverso un aggravio del prelievo, le imprese più forti. Con questi emendamenti, i socialisti propongono una prima misura volta a improntare il sistema di fiscalità d'impresa, non tanto a criteri di redistribuzione interna, quanto a princìpi di premialità ordinaria, intendendo con ciò un abbassamento permanente del prelievo per quelle aziende che realizzino alcune azioni predefinite, portatrici di un effetto sistemico, e tali quindi da realizzare un interesse pubblico. Stanti i ritardi di competitività di cui soffre il sistema produttivo italiano e viste quelle che sono le analisi interpretative di tali ritardi, non ultima quella fornita dalla Commissione Biasco, ci sembra che queste azioni non possano che rientrare nel novero delle scelte che portano una impresa a crescere di dimensioni, ad affrontare investimenti rischiosi per salto tecnologico, a congiungersi col mondo della ricerca, ad aprirsi al mercato dei capitali. Lo stesso Governo ha riconosciuto la validità di una simile logica, adducendo però una mancanza di copertura come motivazione del mancato accoglimento dei nostri emendamenti. Il Gruppo Socialista non intende certo promuovere iniziative prive della necessaria copertura finanziaria, ma non può non sottolineare come la disponibilità di risorse emersa nel corso dell'anno sia stata dispersa in un insieme disparato di spese

Con un apposito ordine del giorno il Governo viene tuttavia impegnato a estendere questo sistema di premialità all'intero territorio nazionale fin dal prossimo anno. A tal fine dovranno essere prioritariamente indirizzati i proventi di ulteriori extragettiti o di altre risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel 2008. Sarà impegno del Gruppo socialista far sì che tale priorità venga puntualmente rispettata, in modo da restituire alla politica per la fiscalità d'impresa la valenza strategica che le è propria.

che il Governo finalmente intervenga per ridurre la pressione fiscale sulle imprese. Ma lo stesso Ministro dell'economia ha precisato che questa manovra sarebbe a costo zero per il bilancio dello Stato, perché attraverso l'allargamento della base imponibile in qualche modo vi sarebbero degli aggiustamenti per i quali alcune aziende sarebbero premiate, mentre altre sarebbero fortemente penalizzate. Intendo affermare che è proprio qui l'inganno. Si sta per costituire un nuovo tesoretto molto consistente, perché complessivamente le aziende verranno fortemente penalizzate da queste misure.

dell'IRES: non sanno che per la stragrande maggioranza delle imprese quel 4,25 significa un importo di imposte di gran lunga superiore all'IRES stessa. Il Governo, Il Governo, con questa finanziaria, gioca sporco, in quanto apparentemente vuol dare la sensazione di ridurre le imposte, la pressione fiscale sulle imprese, ma di fatto la incrementa notevolmente, sottovalutando un aspetto che avevo già sollevato in discussione generale senza ricevere alcuna risposta dal Ministro dell'economia e cioè che le aziende penalizzate sono il cuore del sistema industriale italiano, è già stato detto dal collega Azzolini e da altri, e alle piccole e medie imprese, con questi provvedimenti, verranno tagliate le gambe. tagliate le gambe. Il grido d'allarme è stato lanciato anche da esponenti del Partito Democratico. In discussione generale ho richiamato una lettera mandata al *premier* Prodi

o si porteranno i libri in tribunale oppure si chiuderanno le aziende o si sarà costretti a venderle. E su tutto questo che ho denunciato fortemente durante la discussione generale c'è stata il totale silenzio del ministro Padoa-Schioppa, un segno di grandissima irresponsabilità. Non per nulla ho definito il Ministro non un economista ma un criminale dell'economia*.*

rispetto al risultato operativo lordo, rispetto all'utile cosiddetto civilistico, pagano imposte di gran lunga superiori a quelle che vengono evidenziate, anche dell'80-90 per cento.

serio, sostanziale, in relazione al carico fiscale che sono costrette a sopportare, dichiarano dopo le imposte una perdita di esercizio. Se in questo momento sottovaluterete questa denuncia, vi assumerete la responsabilità

credo che tutti se ne siano resi conto - non vengono più iniziate, né tanto meno concluse, infrastrutture indispensabili non soltanto per mantenere un minimo grado di civiltà e per consentire alle nostre attività produttive

per la prima volta in Italia, ma sicuramente anche in Europa, si comincia ad utilizzare il sistema del *project financing* anche per costruire infrastrutture. In modo particolare le Province di Brescia e di Bergamo hanno raccolto, tra le varie attività industriali, con l'aiuto degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, circa un miliardo e mezzo di euro per la costruzione di 50 chilometri di autostrada che, da Brescia, attraversando la Provincia di Bergamo, arriva alle porte di Milano. Si tratta della famosa Bre.Be.Mi. Cosa succede all'interno di questa finanziaria quando si toccano i temi dell'IRES e dell'IRAP? A fronte di benefici in termini di riduzione di aliquote, si determinano gravi effetti negativi derivanti dalla rimodulazione della base di calcolo IRES che che prevede la sostanziale indeducibilità degli interessi passivi. Proprio in questo caso, i privati che hanno investito un miliardo e mezzo di euro recupereranno tale cifra nel corso di quasi vent'anni di gestione dei pedaggi e nei primi quattro anni di tale gestione, a causa di questa anomalia inserita nel disegno di legge finanziaria, dovranno sborsare circa il 50 per cento di di 60 milioni di euro di interessi passivi non deducibili. Richiamo l'attenzione dell'Aula, dell'opposizione, ma soprattutto della maggioranza, perché vada in porto il primo esperimento dei cittadini, delle attività produttive e delle nostre industrie e che serve per dotarci di quelle infrastrutture che il Governo centrale

la negazione degli ammortamenti accelerati e attraverso l'allungamento della durata dei *leasing* delle locazioni finanziarie e strumentali. Credo

i finanziamenti erogati a queste ultime, a fronte di garanzie prestate da soci qualificati, non venissero dedotti nella misura di un quarto del fatturato aziendale. Oggi, invece, siamo di fronte all'allargamento della base imponibile attraverso l'eliminazione dell'eccedenza degli oneri finanziari nella misura del 30 per cento del margine operativo lordo.

verso il quale andava la *thin cap*; deprime chi vuole rischiare, deprime chi vuole investire, deprime chi vuole intraprendere e vuole far crescere la propria azienda. è una misura inserita in un articolo che è assai gattopardesco, perché è un articolo che tende a far vedere un cambiamento nell'ambito fiscale, ma di fatto non cambia nulla perché rimane sostanzialmente com'è; è iniqua anche perché si distribuisce male tra le imprese; è iniqua perché non mantiene un rapporto tassazione e reddito giusto e lineare. Mi viene in mente l'esempio del fiume dove ad un'altezza di un metro e mezzo qualcuno può annegare, altri rimangono in piedi. Questa è una norma che favorisce le grandi aziende, favorisce le aziende capitalizzate capitalizzate e, rispetto a un tessuto che è l'asse portante vero di questa Nazione e che fondamentalmente soffre di sottocapitalizzazione e di mancanza di investimento, andiamo esattamente nella direzione contraria.

i quali stabiliscono *a priori* il regime di tassazione delle aziende e già in quel caso accade un fenomeno distorto e strano. Ma se anche lo volessimo prendere per buono, abbiamo già stabilito quanto deve ricavare in via presunta quell'azienda, in quel luogo, con quelle strutture. Appesantire ancora quel tipo di aziende - parliamo della piccola azienda - di questa misura iniqua, a mio avviso, è assolutamente sbagliato. Va esattamente nel senso opposto a quello che sostiene il Governo, perché è iniqua, perché tassa lo sviluppo e, tassando lo sviluppo, assolutamente non va verso l'obiettivo del risanamento. I tre pilastri tanto sbandierati dal ministro Padoa-Schioppa sono resi

il possibile scambio tra la salma di Lenin e Diliberto, io proporrei di scambiare invece il nostro vice ministro Visco con la salma di Stalin; mi sembra molto più appropriato. finestra") *(FI)*. Signor Presidente, aggiungerò pochissime considerazioni a quelle già svolte dai miei colleghi con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo che, come è stato sottolineato, costituisce un aspetto tra i più salienti della manovra proposta dal Governo; manovra che è stata annunciata come volta a ridurre significativamente la pressione fiscale sulle nostre imprese e che in realtà - come già è stato dimostrato - nella migliore delle ipotesi ha un saldo nullo, che però per molte imprese si traduce in elementi di incertezza o di appesantimento dell'effettiva pressione fiscale. Comunque, si pone - come ricordava il collega Piccone anche in termini di disincentivo ad una capacità effettiva di capitalizzazione da parte delle piccole imprese. Vorrei soltanto segnalare come ancora una volta queste disposizioni sembrano in parte giustificate dalla scelta tipica del vice ministro Visco di guardare ai comportamenti patologici estremi, ai comportamenti elusivi che in natura sono sempre possibili, per tarare su questi le disposizioni di riforma. Ma è in questo modo che alla fine si costruisce un fisco ostile all'impresa, che comunque non risolve mai per definizione la possibilità di comportamenti elusivi la cui repressione deve essere invece affidata agli organi preposti.

di voler produrre una migliore condizione per quanto riguarda le nostre imprese dal punto di vista

si può preferire alla nuova disciplina quella vecchia ove più favorevole. In questo modo verrebbe salvaguardato l'effetto netto positivo per quanto concerne le imprese. le modifiche introdotte dalla Commissione sono davvero molto marginali. Sono modifiche che hanno certamente qualche profilo qualitativo apprezzabile. Non a caso sono state sollecitate dall'opposizione. Mi riferisco alla compensazione con crediti verso le pubbliche amministrazioni. Ma, dal punto di vista quantitativo, non rappresentano nulla di significativo tanto che ad esse non è stato attribuito un significativo effetto finanziario in termini di minori entrate e, quindi, di minore pressione fiscale sulle imprese.

Ne ha facoltà.

relativo alle opere prime e seconde degli artisti emergenti. Nella precedente finanziaria ci si è fermati esclusivamente alle piccole e medie imprese che poco fanno per gli artisti emergenti e ad

Signor Presidente, con l'emendamento 3.700 si vuole mettere le fondazioni bancarie in grado di disporre di maggiori risorse da offrire al territorio nei settori ammessi, la sanità, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la funzione sociale, l'istruzione e la formazione. Le fondazioni bancarie, lo ricordo, ormai sono diventate protagoniste della nostra società. Sono soggetti privati, autonomi, che operano nel sociale con interventi sempre più qualificati e mirati. La loro creazione, a mio giudizio, è stata una delle più importanti innovazioni istituzionali realizzate nel mondo del *profit*. In questi anni, esse hanno arricchito il nostro Paese con una rete di 88 soggetti, dotati di competenza e autonomia patrimoniale, tutti espressione della società civile. Hanno saputo coniugare le leggi approvate dal Parlamento, che richiedeva loro una graduale riduzione delle loro partecipazioni bancarie e una progressiva diversificazione degli investimenti per tutelare al meglio il patrimonio loro affidato. Hanno migliorato nel tempo la loro capacità di gestione del patrimonio, il che ha consentito di generare cospicue risorse per la loro attività filantropica. In ultimo, hanno fornito una base patrimoniale e finanziaria alla capacità progettuale del terzo settore e di importanti settori innovativi, privati e pubblici, della società italiana, contribuendo a individuare nuove forme di intervento, secondo il principio della sussidiarietà.

ad un prezzo depurato dalle accise. Tale richiesta nasce da una considerazione fondamentale, cioè che la Regione Basilicata

all'estrazione petrolifera, con circa 23 autorizzazioni ed altre 27 per ricerche. Ormai, il 70 per cento del territorio lucano è interessato all'estrazione petrolifera.

canto già in altre parti del nostro Paese, in particolare in Valle d'Aosta e nel Friuli. Dal dibattito che si è sviluppato nei mesi scorsi, sembra che anche il Trentino-Alto Adige stia andando in questa direzione.

è scesa sotto i 600.000 abitanti, questa terra che ha una situazione di crisi aziendale che ogni giorno si evidenzia con chiusure di fabbriche e di aziende, nel momento in cui contribuisce a livello nazionale

La somma prevista per ogni anno è di circa 140 milioni; rispetto ai circa 2 miliardi che lo Stato ricava dalle accise,

che vede una valorizzazione del ruolo delle Regioni nella riscossione dell'IRAP, che costituisce la principale fonte di finanziamento per le amministrazioni regionali, è una valorizzazione che trova fondamento nell'articolo 119 della Costituzione e quindi nel principio di territorialità. Peraltro, ho poi ritrovato l'emendamento riprodotto nel testo della finanziaria. allora: è stato respinto soltanto perché è stato presentato dall'opposizione, pure in presenza di un medesimo contenuto? Era questo tecnicamente possibile? E se non lo era, come penso, constato che veramente ogni giorno si fa un gran parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione (sempre a parole, sempre sulla stampa, finanche ieri e ancora oggi, coerentemente con quella politica degli annunci purtroppo abusata da questa maggioranza), ma poi, quando

dell'IRES, che invece, come loro stessi avranno avuto modo di ascoltare e leggere, le organizzazioni della impresa italiana, Confindustria, le piccole e medie imprese e gli artigiani, hanno formulato un parere complessivamente positivo di questa riforma, evidenziandone talune criticità, che sono state attentamente valutate dalla Commissione durante i lavori

la legislazione vigente prevede, in taluni casi, la indeducibilità assoluta degli interessi relativamente ai meccanismi del *pro rata* patrimoniale e reddituale, mentre questa questa riforma prevede soltanto una diluizione nel tempo della deducibilità degli interessi, che rimangono interamente deducibili. Si è poi proceduto ad alcuni aggiustamenti che riguardano il meccanismo degli ammortamenti per le piccole imprese, eliminando alcuni aspetti di retroattività della disposizione, relativamente agli investimenti già effettuati si è provveduto a precisare meglio la disciplina per quanto riguarda il regime opzionale per le piccole imprese soggette ad IRPEF e ad introdurre, su iniziativa del Governo, questa norma importante della regionalizzazione dell'IRAP, che avvia un percorso di federalismo fiscale vero nel senso di attribuzione alle Regioni, oltre che del gettito di questa imposta anche della possibilità di normare su questa materia. Fatte queste considerazioni, passo ai singoli emendamenti. Il 3.1 prevede la soppressione pressoché integrale della riforma. Quindi il parere è assolutamente contrario,

di progetto: le imprese, cioè, che agiscono per la realizzazione di opere in progetto di finanza possono o no dedurre gli interessi passivi ad esso relativi. Se fosse vera la tesi dei proponenti dell'emendamento, problemi ve ne sarebbero senonché, a mio modo di vedere, questa tesi non è fondata giacché, per la realizzazione delle opere in progetto di finanza è previsto il meccanismo della capitalizzazione degli interessi.

al tema degli interessi; 3.31, considerato anche che relativamente al meccanismo degli interessi vi è stata una norma di chiarificazione introdotta in Commissione relativamente agli investimenti

3.302 affronta il tema della regionalizzazione dell'IRAP, nei termini che ho già detto all'inizio. Francamente, l'ho già detto in Commissione e lo ribadisco, non comprendo

virtuoso, finalizzato ad accrescere i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno e l'onere viene fatto ricadere sul FAS, perché è evidente che una misura di tal genere aiuta lo sviluppo del Mezzogiorno. Esprimo parere

si tende ad eliminare o attenuare il regime sanzionatorio relativo all'eventuale violazione delle norme che riguardano il credito d'imposta per gli studi professionali associati, una misura molto interessante introdotta da questa legge finanziaria. Il parere è contrario

Presidente, vorrei chiedere al relatore, che si è soffermato nell'esprimere parere contrario su molti emendamenti, il perché della sua contrarietà semplice, senza motivazione,

le accise sulla benzina, sul gasolio, sul gas. Una norma, quindi, che sarebbe chiaramente contraria alle indicazioni e alle direttive dell'Unione Europea e creerebbe uno squilibrio difficilmente sostenibile con le altre Regioni.

proprio in questa materia, al ristorno delle accise sulle estrazioni di petrolio alla Regione volto al finanziamento dei progetti di programmazione negoziata. Credo che tale norma costituisca una risposta molto significativa

più che una razionalizzazione costituisce un intervento punitivo e discriminatorio nei confronti, per esempio, del settore del credito contro le banche cooperative e le casse di risparmio

per quanto riguarda l'IRES discrimina le banche cooperative e i piccoli istituti di credito e premia, invece, le grandi banche,

proposta dal Governo è penalizzante nei confronti di quelle imprese che faticano ad innovarsi. Ora, il problema è che noi sappiamo che, tra il 2003 e il 2005, il nostro Paese ha resistito a una vera e propria aggressione da parte del sistema produttivo cinese e indiano grazie ad una profonda innovazione

votare l'emendamento 3.1, che rientra appunto nell'ambito della revisione di questa presunta razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di

Presidente, io le chiedo scusa perché forse lei non è informato che la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza del Senato hanno assunto una deliberazione in merito alla regolarità delle votazioni.

Senatore Boccia, la segnalazione è stata fatta durante la votazione. I colleghi senatori segretari sono intervenuti su mia richiesta nel rispetto del Regolamento cui lei faceva riferimento prima, certificando la regolarità

le argomentazioni fornite dal relatore non mi hanno convinto: è stato molto impreciso ed ha sostenuto che questo emendamento è già nel testo. Non è così. Ritengo che questo intervento legislativo incida profondamente sulla gestione finanziaria delle imprese, in modo particolare per le commesse pubbliche in corso al 1° gennaio 2008. Intendiamo precisare che è invece necessaria una deducibilità per coloro che hanno contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, quelli che soffrono particolarmente i ritardi della pubblica amministrazione. Per questo insisto per la sua

con lo Stato, con le Regioni, con gli enti locali, sono creditrici di somme rilevanti e sono state quindi costrette alle anticipazioni bancarie. È mortificante che, oltre a non poter avere nella patria del diritto ragione in via giudiziaria, dato lo stato di coma profondo del sistema giudiziario civile per cui per una impresa non è possibile ricorrere al tribunale per ottenere soddisfazione, il Governo penalizzi ancor più pesantemente la situazione obbligando le imprese a poter detrarre solo una parte di quelle che sono sue specifiche responsabilità governative. Chiedo la

che cerca di evitare la misura penalizzante per le imprese che ricorrono all'indebitamento e che rischia di limitarne l'operatività.

verso quelle imprese che hanno fatto investimenti in base ai principi normativi di riferimento, che adesso vi accingete a modificare. Siete dei falsari, voi del Governo.

di cui oggi godono le grandi cooperative. Mi riferisco, in particolare, alle cooperative rosse, che sono vere e proprie *holding*, che raccolgono miliardi di euro di risparmi dai propri soci, che in realtà spesso non sono affatto soci, ma semplici risparmiatori, in una condizione di favore rispetto agli imprenditori privati. Quelle grandi cooperative che fanno sognare, tanto per nei confronti delle quali, invece, sarebbe giusto cominciare ad applicare il principio di concorrenza rispetto ai privilegi di cui oggi godono; privilegi anche di recente denunciati nel libro di grande successo Caprotti: «Falce e carrello». Credo quindi che il relatore abbia sbagliato nel rimandare a futura memoria questo intervento perché quando si tratta di libera concorrenza è giusto intervenire immediatamente. Si tratta soltanto di uno dei tanti

l'IRAP è una tassa sul reddito anche quando il reddito non c'è, tant'è che le imprese fanno il calcolo del bilancio normale, calcolano l'utile, a questo utile viene aggiunto il carico di oneri bancari o finanziari più, soprattutto, il monte salari e stipendi, e su questo viene applicata l'IRAP. Sottolineo che quando fu introdotta l'IRAP l'Italia aveva l'11 per cento di disoccupazione e i tassi di interesse più alti di quelli degli ultimi anni: in un momento in cui un Paese in crisi ha tanta disoccupazione e paga forti interessi finanziari, voi avete introdotto una tassa che colpisce gli stipendi e gli interessi finanziari, questo tanto per vedere la lungimiranza di chi governava e purtroppo governa ancora il Paese, ma soprattutto la conoscenza delle cose industriali del Paese stesso. Soprattutto introduce l'obbligo per gli imprenditori, per chi ha delle aziende, di fare falsi in bilancio, perché la questione funziona in questa maniera: un'azienda calcola la base imponibile per il pagamento di tasse come l'IRES; su questo viene calcolata l'IRES; a parte viene calcolata l'IRAP su una base imponibile diversa; l'azienda paga la somma delle due tasse.

ad avere situazioni in cui il carico fiscale sull'utile reale raggiunge l'80-85 per cento, fino addirittura a casi in cui la somma delle due tasse è superiore all'utile. Aziende che teoricamente hanno guadagnato si trovano ad avere debiti verso lo Stato e comunque alla fine ad avere perdite pure in esercizi che teoricamente sarebbero stati in utile. È una cosa veramente incredibile, che solo in un Paese come questo, che lei definisce civile (io un pochino meno

Ovviamente, siamo onesti intellettualmente e sappiamo benissimo che, se nel 2006 avessero vinto la Casa delle Libertà e Berlusconi, l'Europa avrebbe dichiarato illegittima con effetto retroattivo l'IRAP; avete vinto voi, ha vinto Prodi, quindi i suoi amici europei di colpo hanno cambiato idea e l'IRAP è diventata una tassa legittima. Questo però non cambia la sostanza della questione; il nostro resta l'unico Paese in cui si continua ad avere una tassa che di per sé non dovrebbe esistere. Con l'emendamento 3.302 chiediamo che si faccia una cosa logica, cioè che le tasse siano messe in fila

e non come somma delle due tasse. Non ci aspettiamo che l'emendamento possa essere accolto, però rendetevi conto di quello che avete fatto, di quello che continuate a fare e non dovete meravigliarvi se l'IRAP, insieme al canone RAI, è la tassa più odiata dagli italiani. Dobbiamo poi aggiungere

aprire un dibattito, anche se breve, sulla politica di tipo assistenziale portata avanti dal Governo

del Governo, anzi all'inasprimento di alcune misure nei confronti di quella piccola e media industria che - vorrei ricordarlo agli amici della Lega

che va a colpire gli interessi - sarebbe sbagliato colpire gli interessi - e che va a scrutare che cosa succede nell'industria di Stato,

si autorizzano investimenti nei confronti della grande impresa, non pensando che invece esiste una piccola e media industria che in questo momento soffre sia al Sud che al Nord Italia. L'IRAP è quella tassa malefica

non pensò a quanto la piccola e media industria realizza in termini di PIL non soltanto a Varese ma anche a Catania e a Palermo.

Avete votato contro l'emendamento che sosteneva la destinazione di 200 milioni di euro al Fondo di rotazione garantito e gestito dal Ministero a favore della piccola e media industria in Sicilia.

Noi diciamo che questa è la maggioranza dei salotti buoni, *radical chic*, dei cappottini, dei pullover di cachemire, dei consigli di amministrazione

tenere presente anche un milione e mezzo di piccole industrie, di artigiani, di piccoli imprenditori. A questi la Casa delle Libertà

Riteniamo di dover incidere in qualche modo attraverso una modifica legislativa che tenga conto anche di questo aspetto. Pertanto, ribadisco l'importanza dell'emendamento

scomparsa. Mi auguro che ci sia un sussulto in questo senso anche da parte di coloro che in Commissione finanze ne condividevano lo spirito. Chiedo

a denunziare quello che avviene in questo Paese. Questo è un Paese in cui il Governo fa dichiarazioni in Aula per cui la copertura non c'è, ma comunque le risorse ci sono nella buona sostanza; in cui una

che è ingiusta e che non dice quello che avviene in questo Paese, un Paese in cui la pressione fiscale è aumentata dal 40,6 a più del 43 per cento durante questo esercizio finanziario. Chiediamo al Parlamento di votare a favore del nostro emendamento 3.63 e contro questo Governo.

Presidente, l'emendamento 3.64 limita gli effetti perversi di queste misure: l'IRAP, che si è voluta diminuire dal 4,25 al 3,9 per cento in relazione all'allargamento della base imponibile, può raggiungere percentuali incredibili rispetto al risultato operativo lordo, cioè all'utile civilistico.

che per la loro base imponibile, per taluni costi indeducibili - immaginate le società di servizi, che fanno ricorso ad automobili, a

per non penalizzare molte piccole e medie imprese. Su

Come hanno già dichiarato in precedenza nell'illustrazione i senatori Azzollini e Sacconi, l'emendamento 3.66, presentato da noi insieme agli amici della Casa delle libertà, consente ai contribuenti, in particolare alle imprese, in questo momento per loro così difficile, di applicare nella propria dichiarazione dei redditi le norme a loro più favorevoli. Ciò viene richiesto in quanto le norme fiscali e tributarie, presentate in questa finanziaria, sono peggiorative rispetto a quelle degli anni precedenti.

le categorie dell'imprenditoria minore. Collega Legnini, lei ha detto di aver trovato l'accordo di tutte le organizzazioni degli

abbiamo avuto tutt'altra opinione. Si sono dichiarate molto preoccupate perché, mentre con una mano operavate la riduzione dell'IRES

Non è vero! Smentite voi essi perché nella relazione tecnica del Governo è scritto che questa manovra comporterà una maggiore entrata

avrà un aggravio di pressione fiscale. Voi non sapete nemmeno mentire perché avreste almeno dovuto non scrivere nella relazione tecnica l'esatto opposto di quello che dite.

in questa chiave. Non possiamo continuare a trattare il contribuente come un povero soggetto da vessare; quel minimo rispetto dei diritti e della dignità della persona e della libertà individuale e di impresa dobbiamo poterla garantire, anche in nome di quel codice che ci siamo dati, ma che continuiamo a non applicare, che difende

Il relatore e il Governo hanno ravvisato una sostanziale concordia con la nostra proposta, ma hanno ritenuto eccessivamente oneroso il ripristino della norma della scorsa scorsa finanziaria. La quantità di soldi spesi per altro potrebbe tranquillamente giustificare uno sforzo per ricondurre la questione dei crediti d'imposta vanificati per le imprese ad una sua più razionale sistemazione. Se entro il termine del dibattito in Aula i senatori e il Governo vorranno rivedere la loro posizione, ciò sarebbe utile per migliaia di imprese che si trovano di fronte questa norma, che, ribadisco, è retroattiva e particolarmente onerosa per le imprese che vi avevano confidato.

Presidente, il Gruppo socialista ha presentato una serie di emendamenti che tendono a recuperare il fisco come strumento di politica economica che orienti il Paese alla crescita e alla competitività, quindi cercando di favorire, attraverso una fiscalità premiale, le azioni virtuose delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, si collegano ai mercati finanziari, che compiono crescita dimensionale. Ci è stata addotta dal Governo una mancanza di copertura. Noi ne abbiamo preso atto, anche se rileviamo ovviamente, essendo all'indomani dell'approvazione del decreto, che nel decreto sull'extragettito molte risorse sono state sprecate in mille rivoli invece che in interventi strutturali. Abbiamo comunque accettato la riformulazione del Governo che, con un inizio di impegno in termini di risorse, anticipa in alcune aree del Paese questa fiscalità premiale e, con un ordine del giorno successivo, profila un impegno forte perché questo metodo venga in via definitiva poi allargato al resto del Paese. Riteniamo molto importante questa strumentazione fiscale perché anche attraverso il fisco si può ridare qualità, crescita e competitività al sistema produttivo italiano.

Presidente, provvidenzialmente, vi è l'emendamento 3.86 che riguarda esattamente l'*ex* comma 18 che, nella versione licenziata dalla Commissione, è il comma 23 ed è esattamente quello

consentito a degli imprenditori del Mezzogiorno, che avevano diritto al credito d'imposta, di poterlo utilizzare per gli anni 2007 e 2008. Gli imprenditori, sulla base della norma dell'anno scorso, hanno utilizzato il credito d'imposta nel 2007; siamo già a novembre e, quindi, quasi tutti lo hanno fatto, impostando la loro politica di bilancio per il 2008 con l'utilizzo di tale credito. Inopinatamente, il Parlamento quest'anno cancella la norma della finanziaria dell'anno scorso. Mi consenta un'osservazione che ho già fatto in altre occasioni: ormai, quando in Italia approviamo una norma, è già tanto se dura un anno. Come è noto, infatti, questa finanziaria si esercita a cancellare molte norme della finanziaria dell'anno scorso, ma in questo caso, si commette un errore, perché gli imprenditori avevano già progettato la loro politica d'investimento sulla base della norma Il danno è oggi notevole per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno perché l'utilizzo è stato già realizzato; ciò significa non poter utilizzare più il credito d'imposta e restituire quello già utilizzato sulla base di una norma retroattiva.

qualsiasi investitore e, ribadisco, la fiducia dell'investitore nella certezza delle norme è fondamentale: togliergli una norma sulla quale ha fatto affidamento è gravissimo, sarà indotto a non investire più. Questo è il senso dell'emendamento Ho chiesto più volte al Governo ed alla maggioranza di ripensarci; francamente, sul piano intellettuale hanno riconosciuto la validità delle nostre obiezioni, mi si dice però

il migliore degli aspetti di cui tener conto, esattamente si colpiscono ancora gli investimenti.

davvero nello sconcerto le imprese che in Italia, ogni giorno, sulla fiducia di norme esistenti, provano a fare andar avanti questo Paese.

Colleghi, prendete posto, per cortesia, capisco la stanchezza, ma abbiamo ancora un'ora e mezzo di lavoro prima dell'interruzione dei nostri

nel senso che quando lunedì abbiamo ascoltato la sicurezza del Ministro dell'economia sapevamo che non c'era la copertura per l'emendamento presentato in Commissione. Forti di tale convinzione, abbiamo presentato un emendamento che riguardava i *ticket*,

Il Ministro dell'economia, che ha voluto fare una disputa accademica con il Ragioniere generale dello Stato, è uscito sconfitto e umiliato dalla presentazione di un nuovo emendamento che ha cancellato la precedente soluzione. Signor Presidente,

preannuncio il voto contrario a questo emendamento per una questione di armonia di tutto l'impianto della legge finanziaria

è centrale proprio per lo sviluppo che la legge stessa, accanto al al problema della stabilità e della perequazione sociale, porta avanti.

forse tutto l'effetto di questa manovra organica. Vorrei ancora ricordare

svolgere una brevissima dichiarazione di voto semplicemente per invitare i colleghi ad esaminare un problema di equità di tassazione su terreni fabbricabili

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo emendamento. Non comprendo le tante parole che questa maggioranza esprime riguardo ai giovani, specialmente nel campo dell'aiuto agli artisti emergenti. Qui parliamo di produzioni musicali, di aiutare le società che

Altro che parlare dei *festival* di Roma e dei tanti altri che servono solamente a tagliare nastri e a passeggiare con le attrici. Qui non si fa altro che mettere in un angolo i giovani che vorrebbero artisticamente progredire. *(Applausi

senatore Caruso. Non preciso di graduare il vantaggio fiscale per le aggregazioni che si formano in funzione che alle stesse potessero partecipare dei giovani professionisti. Questi emendamenti non sono stati considerati in Commissione bilancio e dal Governo e me ne dispiace. Sono d'accordo con lei, signor Presidente, quando a chiosa di un intervento del senatore Paravia ha inteso affermare che questo è un Paese civile; sono anche molto d'accordo tuttavia con il senatore Paravia quando egli ha inteso osservare che questo Paese si comporta in maniera incivile quando cambia le regole del gioco mentre il gioco è in corso e - aggiungo io - quando non sostiene il proprio futuro e le proprie generazioni. In questo senso, non solo è un Paese poco civile, ma anche un Paese stupido perché perde di credibilità nell'una e nell'altra occasione. Invito il relatore, di cui conosco il valore,

Il senatore Legnini ha sostenuto che volessi attenuare la portata delle disposizioni togliendo la sanzione che viene indicata in alcuni di questi commi. Non è così, senatore Legnini, io ho inteso fare un'operazione diversa. Posto che il Governo non ha precisato di quale sanzione si tratti, quindi può essere una sanzione amministrativa, una sanzione fiscale, ma anche una sanzione penale, ho inteso sottrarre alla disponibilità del Governo di provvedere con un semplice decreto interministeriale a stabilire delle sanzioni. Credo, senatore Legnini,

Ritiro infine l'emendamento 3.107, signor Presidente, che è stato riscritto - non da me - per adattarlo alla nuova numerazione del testo ma non è più attuale. più attuale. Si è verificato un miracolo legislativo, nel senso che la proposta che avevo presentato alla Commissione bilancio, che mirava a togliere la tautologia che esisteva

non è stato approvato, ma ne è stata approvata in maniera misteriosa l'intenzione. Il senatore Morando ci ha spiegato che dovremmo modificare alcune norme del nostro Regolamento, a me piace dirgli che sarebbe bene controllasse che il Regolamento venga applicato puntualmente nella sua Commissione.

Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.106, appena illustrato dal senatore Caruso. Non si tratta di stabilire la civiltà di un popolo, ma la modernità e la coerenza dei propri comportamenti. Nella riforma delle professioni alcune delle cose sostenute dal ministro Bersani sono state considerate positive e altre no, ma ce ne sono alcune che hanno un grande significato: allargare e modernizzare il rapporto all'interno delle attività professionali dilatando la platea dei compartecipi, specialmente i giovani. Sono un vecchio avvocato e non nascondo che tra i difetti della categoria - e ne ha molti - c'è anche quello di avere nei confronti dei giovani un atteggiamento paternalistico: vengono utilizzati e poi gettati quando non servono più perché diventano concorrenti. E' bene invece allargare il rapporto, far sì che i giovani diventino partecipi della vita di uno studio legale o di uno studio professionale in genere, acquisire queste forze nuove in funzione del loro futuro. Vogliamo chiuderci nella visione esclusivista dello scagno chiuso solo da parte dei super-iniziati e dei super-professionisti, vogliamo invece vedere se la società ha bisogno anche di altri soggetti, di altre forze e di altre speranze? Perché la libertà della professione è la garanzia dei cittadini, e solo se il professionista è libero anche economicamente può svolgere quella funzione di tramite tra l'interesse privato e l'esigenza pubblica di rendere ciò che è privato corrispondente alle esigenze della collettività. Ecco perché sono onorato di aggiungere la mia firma all'emendamento del senatore Caruso e credo che sia una cosa che dovrebbe unirci, cari amici e cari colleghi anche di cosiddetta controparte. Non considero il Parlamento una parte ed una controparte, considero un'area nella quale il consenso e il dissenso si formano liberamente e si formano sulla base dell'intelligenza e della comprensione anche delle ragioni degli altri. Se non ce la fate a fare questo, anche in questo caso, non venite a dire poi che siete moderni: siete conservatori e antiquati.

a stare attenti ad alcune espressioni che usiamo. Tutti quanti noi rappresentiamo qui il popolo italiano e siamo espressione della sovranità popolare,

Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le osservazioni fatte dal senatore Caruso e poi dal senatore Biondi. In realtà, l'emendamento sopprime il potere in capo al Governo di determinare con decreto ministeriale le sanzioni, ove le condizioni richieste per l'accesso al credito d'imposta relative alla costituzione degli studi professionali associati venga meno. È evidente che l'accoglimento di questo emendamento, di cui comprendo le ragioni e il valore, determinerebbe il venir meno di qualunque sanzione per il caso, appunto, nel quale i giovani professionisti associati, o i meno giovani, violassero le regole che sovrintendono alla concessione di questo beneficio, in particolare la sensibile riduzione

per le Regioni Basilicata e Campania, soprattutto nel settore creditizio, a seguito del succedersi degli eventi calamitosi. È stato previsto che il prolungamento sino all'anno 2010 avrebbe completato definitivamente il quadro ricostruttivo sia per la Basilicata che per la Campania

Presidente, vorrei sollecitare il Parlamento a riflettere su questo voto, che interviene su una misura specifica indispensabile a un sostegno minimo all'impresa all'impresa siciliana, ma anche della Valle d'Aosta, perché è una norma che riguarda il finanziamento degli investimenti in queste due Regioni a Statuto speciale e che per la Regione siciliana assume caratteri surreali. l'esiguità del finanziamento, soli 40 milioni di euro, ha determinato il fatto unico che il bando del Ministero dello sviluppo economico, aperto in data 22 novembre 2006, è stato richiuso nella medesima giornata dato il numero elevatissimo di istanze - circa 1.500 - di imprese che hanno ritenuto di poter accedere, alla luce dei requisiti previsti dalla legge, a questo tipo di finanziamento. Ebbene, per il regolamento applicativo di questa normativa, se la norma non viene finanziata in modo congruo (io chiedo un intervento integrativo di 200 milioni di euro, che è una misura ragionevole per un investimento di questo tipo), butteremo risorse. oltre ad una difficoltà gestionale degli uffici a corrispondere in tempi ragionevoli queste risorse, per il meccanismo che prevede che prevede una suddivisione omogenea delle risorse a tutte le aziende che hanno fatto istanza, rispetto alla possibilità di un credito d'imposta che può pervenire sino al 50 per cento per l'acquisto di macchine utensili, avremmo un risultato massimo dell'8 per cento. Voi capite che un credito d'imposta dell'8 per cento sull'investimento in infrastrutture e macchinari è francamente ridicolo. del disegno di legge finanziaria, che è stato tanto evocato come uno strumento di sostegno all'impresa, certamente ha contenuti importanti, probabilmente patteggiati con la grande industria di Stato, ma ha perduto un'occasione, quella di contenere al suo interno misure agevolative differenziate per le aree del Mezzogiorno, quanto meno quelle ad obiettivo convergenza, che hanno bisogno di un differenziale significativo rispetto ai meccanismi di incentivazione, meglio ancora se incentivazioni automatiche, senza mediazioni né politiche, né professionali, perché questo che è ormai un *leitmotiv* degli ultimi residui di politica meridionalista, che vede soltanto nella fiscalità compensativa o di vantaggio uno strumento strutturale per innestare processi di sviluppo, da questa manovra finanziaria viene completamente disatteso. La mia proposta è minimale, non ha la pretesa di una modifica strutturale del sistema degli incentivi o delle agevolazioni. C'è un mio emendamento molto più ambizioso, oserei dire velleitario, che prevede un intervento ampio e strutturale, ma questa è una misura minima, che viene tra l'altro dagli ambienti imprenditoriali, assolutamente *bipartisan*, che avrebbe preteso quanto meno dal relatore, dalla maggioranza e dal Governo un'attenzione intellettualmente un po' meno pigra.

presentati all'articolato di questa finanziaria che apre una discussione sul Mezzogiorno. Il Governo ha

affermando che le risorse rese disponibili per il Mezzogiorno negli anni a venire da questo Governo non hanno paragoni e presentando all'Aula una decisione di intervento per 100 miliardi di euro. Anche qui, mi sia permesso, siamo di fronte che si possono riferire all'abitudine di questo Governo al «si dice, ma non si fa», perché il Governo dice che sono disponibili per il Mezzogiorno 100 miliardi di euro e invece questa disponibilità nei fatti non esiste, è una falsità, e cercherò di dimostrarlo nell'ambito della mia dichiarazione di voto a favore dell'emendamento del senatore Pistorio.

di un intervento espropriativo nei confronti delle competenze che erano state appostate a favore del Mezzogiorno. Ma il Governo come mistifica i dati? Dichiara: è vero che abbiamo diminuito il Fondo per le aree sottoutilizzate, ma stiamo prevedendo, come contributo italiano al bilancio europeo per europeo per le risorse destinate alle aree coperte dalle iniziative plurifondo, quindi per il periodo 2008-2010, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quella precedente.

perché quella è una competenza che, come è successo per i programmi precedenti, viene ad essere utilizzata verso la fine attuativa del programma europeo: quindi, se quest'ultimo parte dal 2008, ciò significa che quella cifra, appostata per gli anni 2008-2010,

sostanza», e non per una copertura, ma per una disponibilità che nella buona sostanza non esiste, perché dire che si provvede alla competenza per i programmi europei plurifondo

Presidente Angius, credo che un Paese veramente civile dovrebbe avere un residuo fiscale pari a zero. Ebbene, il residuo fiscale nelle Regioni del Nord è di 100 miliardi ogni anno.

Noi siamo d'accordo sull'esigenza di affrontare, in un'ottica di coesione nazionale, il tema del federalismo fiscale, perché siamo consapevoli che bisogna investire, soprattutto nel Sud, nella cultura della responsabilità. Ed io intervengo non tanto per sostenere il dato quantitativo presente all'interno dell'emendamento che pur voteremo come Gruppo di Alleanza Nazionale, ma per sottolineare in termini politici la straordinaria contraddizione della maggioranza,

importante per sottolineare una contraddizione politica del centro-sinistra, che contraddice l'impianto della finanziaria votando emendamenti che utilizzano la leva fiscale a fini di politica economica. allora: se così è, perché avete utilizzato l'alibi della copertura quando avete utilizzato il FAS per il credito di imposta per le assunzioni? Non potevate utilizzare il FAS ai fini di politica economica, cercando di far approvare i due emendamenti che voi stessi avete presentato? Il problema, Presidente,

il problema è il sistema di potere meridionale del centro-sinistra che utilizza le risorse a fini di clientela e di frantumazione degli interventi! Caro Castelli, siamo d'accordo: è un problema politico, non quantitativo. La sfida che tutto il centro-destra deve raccogliere in nome del Nord e del Sud è una sfida politica, non una sfida di contrapposizione che non c'è. Tutto il centro-destra della responsabilità e della stessa cultura dello sviluppo e dell'investimento nelle grandi risorse che il Mezzogiorno deve sviluppare in termini di cultura autopropulsiva, liberando la società meridionale dalla compressione della casta politica e del sistema di potere, da Vendola a Bassolino!

questo emendamento ci dà la possibilità, sia pur brevemente, di dialogare sul tema. Sarebbe molto semplice - lo dico rivolgendomi ricordare come per cinque anni, nella passata legislatura, chi ha governato questo Paese abbia sostanzialmente subito il pesante veto di alcuni partiti di maggioranza su scelte per il Mezzogiorno di cui il Paese intero aveva bisogno. Ora ci troviamo davanti ad un Governo che già nella finanziaria per il 2007, e ancora di più - e lo dimostrerò tra poco - nella finanziaria per il 2008 ha assunto importanti decisioni per il Mezzogiorno, per il Mezzogiorno, proprio scegliendo l'impostazione degli automatismi contro quella discrezionalità dei sostegni che, attraverso una certa intermediazione impropria, ha rischiato spesso di vanificare l'efficacia degli interventi. Chiedo con molta semplicità e molta chiarezza: l'abbattimento del costo del lavoro, il cuneo fiscale, esisteva prima? Il credito d'imposta sugli investimenti, che sta per diventare realmente operativo, era stato introdotto prima? Il coraggio di ripristinare il credito d'imposta sull'occupazione, che in passato è servito a combattere il lavoro nero e ad incentivare l'occupazione del Sud, vi era prima? Lo dico ai colleghi meridionali del centro-destra. Rispondetemi: c'erano prima questi provvedimenti? Viespoli, hai avuto il coraggio di assumere come centro-destra questi provvedimenti nella passata legislatura? legislatura? I 30.000 *stage* per i giovani laureati del Mezzogiorno c'erano prima

Altro è la comunicazione, di come si sanno presentare al Paese alcune scelte. Posso anche essere d'accordo che c'è un *deficit*. Posso anche convenire che la scelta saggia che il Governo ha adottato di unificare il FAS, i fondi europei, la spesa ordinaria in unica possibilità di spesa che consente una programmazione più facile, ha bisogno di una progettualità organica per i prossimi anni. Questo è vero. Lo dico da tempo e da tempo ho chiesto al Governo che la programmazione, il progetto organico sul Mezzogiorno ci sia. Su questo dobbiamo spingere tutti quanti. Ma negare che nella finanziaria dello scorso anno ed in questa ci siano scelte chiare a favore del Mezzogiorno, che eliminino quella pericolosa discrezionalità e che rendano automatici i sostegni,

gioiosa concretezza e coerenza di avere innervato un processo virtuoso che potrà, con una risposta dal basso che verrà dalle Regioni meridionali, pian piano concorrere a farci uscire da questa *impasse*.

tant'è vero che ieri ho votato in contrasto con il mio Gruppo persino gli emendamenti del senatore Turigliatto, che poi ha votato contro le politiche a sostegno delle famiglie.

rientra nel Sud, nel Mezzogiorno o è collocata al Nord. È un problema di geografia, non solo politica. Nel dicembre 2001 la Campania, con una delibera CIPE, ha ottenuto dal Governo Berlusconi 18.000 miliardi di lire. Sostenere, di fronte a questi stanziamenti ed a queste enormi risorse affluite in Campania, che il Governo Berlusconi per il Sud non ha realizzato assolutamente nulla

affermò che la giunta Rastrelli aveva radicalmente invertito il percorso della Regione Campania. Infatti, la Campania non utilizzava i fondi comunitari

basta pensare alle grandi infrastrutture che furono realizzate in quel periodo. Il senatore Viespoli, come sottosegretario al lavoro, pose in essere delle politiche di di intervento sul lavoro e sulla professionalizzazione dei disoccupati, che poi furono disattese dalla Regione e dalla Provincia di Napoli, che trasformarono il tutto in un voto di scambio e clientelare con alcuni settori dei senza lavoro. Questa è la realtà. Sento qui alcuni colleghi dire che il centro-destra non ha realizzato nulla nel Mezzogiorno, non ha speso una lira; sono menzogne smentibili anche a livello macroeconomico.

che è. Condividiamo la proposta del senatore Pistorio perché lo Stato deve rispettare le norme sulla finanza siciliana, una finanza che è prevista da uno Statuto speciale, quindi c'è un'autonomia che va rispettata, non violata. Dallo scorso anno abbiamo assistito ad una distorsione e ad un mancato rispetto di queste norme. Non occorrerebbe una legge per far rispettare tutto ciò, trattandosi di un momento importante nei rapporti tra Regione Sicilia e Stato. Ma veniamo al punto. L'onorevole Pistorio pone una questione di grande rilievo: il rispetto dei finanziamenti che derivano dalla ex legge Sabatini. Ebbene, la legge Sabatini è stata la più grande e la più straordinaria legge di sviluppo di questo Paese. Ha determinato la crescita delle piccole e medie imprese, l'innovazione tecnologica, la responsabilità delle banche rispetto ad un'alimentazione della domanda

nel momento in cui essa è impegnata in uno sforzo di adeguamento. Noi invece vogliamo uno sviluppo non duale, uno sviluppo unitario. Caro senatore Castelli, soltanto dallo sviluppo del Mezzogiorno far scaturire una crescita dell'intero Paese, una crescita che porti benefici soprattutto al Nord, perché è di questo che ha bisogno quel mercato per poter diffondere le proprie merci. Per queste ragioni, Presidente, credo che l'onorevole Bersani, Ministro dello sviluppo economico, abbia fatto un grandissimo errore quando ha costituito quel fondo distruggendo

l'emendamento pone una questione assolutamente delicata e chiedo che l'Aula responsabilmente valuti l'importanza della questione che sta dietro l'emendamento 3.700. Con il senatore Grillo ho condiviso molte battaglie in passato ma in questo caso ho qualche dubbio e perplessità.

in particolare le fondazioni bancarie. Io mi sono permesso di mutare questa espressione in «foresta partecipata», nel senso che partecipano a tutto ma diventano sempre più impenetrabili. *(Applausi dal Gruppo

Si è tentato persino di farle partecipare al capitale delle banche popolari determinando le condizioni per un loro asservimento. Ma oggi non è così: noi dobbiamo fare chiarezza su questo, non possiamo consentire che ci sia un simile regalo. Onorevole Rossi, onorevole Turigliatto, nei giorni scorsi vi siete impegnati sui problemi bancari, anche ieri sul problema dei mutui, ma il prodigio di questa maggioranza è avere costruito una Repubblica bancocentrica con un triangolo tra il tesoro e le grandi aziende bancarie. Questo è quello che noi denunciamo e i regali che ci sono in questa finanziaria lo stanno dimostrando. I fondi di investimento rispondono a qualcuno, rispondono dei loro risultati,

Signor Presidente, sono veramente sorpreso che il mio collega e amico Eufemi abbia preso una cantonata così enorme.

dibattito è datato, collega Eufemi: 15 anni fa qualcuno si permise di dire che le fondazioni bancarie erano enti autoreferenziali, in realtà, le fondazioni sono diventate protagoniste positive della vita civile, sociale ed economica del Paese.

Insisto perché l'emendamento venga accantonato. Voglio spiegare al collega Eufemi che in questo caso non viene addebitato alcunché allo Stato; si tratta semmai di dare meno tasse allo Stato e consentire che queste minori tasse che vengono versate al Governo centrale le abbiano le fondazioni in dote per intervenire in tutte le Province del nostro Paese in una logica, questa sì, davvero federale.

che obbliga le aziende del turismo e le agenzie di viaggio a fornire l'elenco clienti; cosa che non è mai stata messa in atto né dal precedente Governo di centro-sinistra, né, tanto meno, quando è stato abolito complessivamente l'obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori. Chiediamo

io non giudico positivamente questo articolo per la semplice ragione che, ancora una volta, si interviene, abbastanza significativamente, a favore delle aziende riducendo fortemente le aliquote.

consonanza o disponibilità ad intervenire in senso largamente più positivo a favore di questi settori sociali. Ancora una volta, è una immediata disponibilità rispetto a quelli che io considero settori privilegiati della società, in questo caso le aziende, con una riduzione ulteriore delle aliquote.

in riferimento alla parte dell'articolo che rimodula da un lato l'aliquota IRES e, dall'altro, la base imponibile, che questo articolo produrrà un incremento della pressione fiscale. Produrrà quindi, perché non è riconosciuto nelle cifre di bilancio, un maggiore introito

sostiene che questa finanziaria non crea un incremento fiscale. Purtroppo, poi, la rimodulazione delle aliquote della base imponibile creerà una redistribuzione del carico fiscale all'interno della platea delle imprese soggette all'IRES a favore della grande impresa e a sfavore della piccola e media impresa. Senza entrare nel merito

ben impiegato come maschera per nascondere una maggiore imposizione fiscale. Tanto è che, come a tutti noto, questa finanziaria creerà, oltre ad una

pressione fiscale e del maggiore indebitamento dell'esercizio 2008 non ci saranno risultati positivi per il Paese. Questa, quindi, è la motivazione concreta, seria.

con l'altra mano aumentando la base imponibile. Talché, il risultato netto per il sistema delle imprese è nullo, perché si abbassano le aliquote da una parte e si aumenta la base imponibile dall'altra. Per il sistema delle imprese, complessivamente, non c'è un'azione di sviluppo. È vero che all'interno del sistema stesso, poi, si determina anche una distribuzione sperequata a vantaggio delle grandi imprese, a danno di quelle piccole e di quelle più indebitate: è un meccanismo che anziché guardare alla produttività e alla competitività delle imprese, guarda alla consistenza del capitale. Vorrei poter dire che è un testo capitalistico, capitalistico, se per me questa non fosse una valutazione positiva, anziché negativa. Ma il risultato è che determina agevolazioni ad alcuni grandi che possono autofinanziarsi e andare magari sul mercato con emissioni, ma svantaggia quelli che hanno idee innovative, competono di più, hanno ammortamenti accelerati perché sono più tecnologizzati: in sostanza, sono le imprese che dovrebbero essere più orientate all'esportazione. È dunque un meccanismo miope,

di più la tassazione sulle imprese e non hanno aumentato la base imponibile: le imprese tedesche sono quindi più competitive di quelle italiane, pur essendo in un contesto di economia

netto, un effetto di sviluppo sul sistema imprenditoriale. Si sostiene che non ci sono le risorse. Non è vero, signor Presidente, perché la maggioranza avrebbe ben potuto evitare quei miliardi di euro di spese clientelari disposti da questa finanziaria sulla base degli emendamenti approvati in Commissione. Se si fosse comportata correttamente in questo senso, avrebbe trovato le risorse per operare una riduzione netta della imposizione sulle imprese. nella *voluptas* di accontentare tutti per cercare di salvaguardare in qualche modo un consenso (azione che sappiamo comunque che non le servirà), ha rinunciato a fare con questa finanziaria quell'una o due azioni incisive che si sarebbero potute fare: avrebbe potuto limitarsi seriamente la tassazione per le imprese; avrebbe potuto limitarsi ad aumentare il reddito per gli strati più deboli della popolazione; non ha fatto né questo né quello e non si è neppure limitata, questa volta, nello spendere e spandere per accontentare le proprie clientele. La cosa non va assolutamente bene.

all'articolo 3, che rappresenta in modo emblematico l'atteggiamento di questo Governo in tutti i suoi comportamenti, caratterizzato da una connotazione da una connotazione fortemente ideologica nelle proprie scelte e da una connotazione di totale mistificazione nel comunicare all'Assemblea e al Paese le decisioni vere che sta assumendo. Farò solo tre esempi,

da una parte, con una riduzione forte di pressione fiscale per grandi imprese, banche e assicurazioni e, dall'altra parte, da un enorme aumento di pressione fiscale per le piccole e medie imprese. Su tutti emerge il caso dell'IRES:

della politica politicante, della politica delle clientele, che i contribuenti pagano con maggiori tasse e meno servizi: meno cittadini ma più sudditi. In terzo

anno. Vorrei che si prestasse maggiore attenzione a tale questione, perché abbiamo il dovere, soprattutto nei confronti di una Regione piccola, che probabilmente ha poca possibilità di essere sostenuta da un considerevole numero di rappresentanti del Parlamento, di verificare se le obiezioni poste dal relatore hanno un fondamento. Il relatore parla dei vincoli, e nell'emendamento presentato

da parte dei presentatori, di non voler andare avanti come carri armati, ma di approvare una norma che consenta poi di intavolare una discussione seria rispetto ai vincoli esistenti. Un'altra questione è legata all'avvenuta modificazione del quadro normativo. Vede, relatore, io ho vissuto anche un'esperienza amministrativa di importante livello e ricordo le discussioni - lo ricorderà anche il senatore Ghigo con l'allora Presidente della Regione Basilicata, il senatore Bubbico, il quale sollevava con le Regioni il tema dei proventi da restituire ai cittadini della Basilicata per quanto riguarda la produzione di petrolio,

Ho partecipato, nelle settimane scorse - lo dico al relatore e spero di trovare la sua attenzione - ad un'assemblea di amministratori dell'una e dell'altra parte politica (ero in giro per la Regione per presentare il mio nuovo movimento),

di non essere intervenuto su questa materia. Oggi scopriamo dal relatore che nella finanziaria del Governo Berlusconi un emendamento avrebbe risolto questa materia. Evidentemente, o non è vero o nessuno ne è a conoscenza o non ha prodotto effetti sulla legislazione in favore di quella terra.

c'è un diritto al ristoro per i cittadini di quella terra. Questo è il tema che pone l'emendamento, è un tema che si pone come fondamento normativo e che poi avrà seguito amministrativo nell'attuazione della stessa norma. Credo che sarebbe una cattiveria verso la Basilicata negare il diritto d'accesso nella legislazione italiana a questo emendamento. Lo dico soprattutto perché in quest'Aula oggi, come sempre del resto, ed è una presenza frequente, c'è il presidente Colombo che ha dimostrato

in questo caso sarebbe opportuno partecipare, evitando che prevalga una logica d'appartenenza contrastante con gli interessi della Basilicata. finestra"). Informo i colleghi che è arrivata una brutta notizia. Pochi minuti fa, un elicottero statunitense decollato dalla base di Aviano è precipitato presso Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. A bordo c'erano 11 persone. Sono in corso verifiche ed accertamenti su questo disastro;

terra che ormai si avvia a fornire il 25 per cento del petrolio nazionale. Inoltre, vorrei ribadire al senatore Legnini che nella finanziaria dell'anno scorso ha confuso un problema di *royalty* con un problema di accise.

verso fondata, tuttavia (come ho detto ai colleghi, oltre che amici, con i quali ovviamente non posso che condividere una battaglia a favore della nostra terra)